L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente, alla luce dell'andamento dei lavori della 5a Commissione permanente sul decreto-legge PNRR e politiche di coesione. L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione del decreto-legge sulla cessione dei crediti di imposta, approvato dalla Camera dei deputati, anche ove non concluso dalla Commissione. I tempi della discussione generale sono stati definiti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Poiché il Governo ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto. L'esame del provvedimento potrà concludersi nella seduta di oggi, che non prevede orario di chiusura, o proseguire nella mattinata di domani. La prossima settimana i lavori dell'Assemblea riprenderanno mercoledì 12, alle ore 15, con la discussione della mozione a firma dei senatori Boccia, Floridia Barbara, Paita, Unterberger e De Cristofaro sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Seguirà l'esame del decreto-legge PNRR e politiche di coesione, con sedute fino a venerdì 14 aprile, ove necessario. Restano fermi gli altri argomenti già previsti dal calendario dei lavori approvato il 21 marzo.

sostenere la proposta fatta dalla maggioranza e dal Governo sul calendario. Il Partito Democratico non ha condiviso tali proposte perché esse, signor Presidente, cancellano con un tratto di penna lo sforzo che tutti noi stiamo facendo nelle Commissioni per provare a dare un senso al nostro lavoro. Lo dico perché in questa settimana avremmo dovuto lavorare su due provvedimenti, prima di tutto nelle Commissioni,

abbiamo più volte sottolineato anche in Conferenza dei Capigruppo - è una vera e propria manovra. Come lei sa, signor Presidente, i pareri sono arrivati solo ieri sera, dopo lunghe giornate di attesa,

all'improvviso la maggioranza ha deciso di assumersi la responsabilità di smontare e rimontare una *governance* che aveva già caratterizzato una serie di discussioni nei due rami del Parlamento. Ma il tema di fondo è che noi chiedevamo più tempo per approfondire alcuni aspetti che incideranno in maniera evidente su temi che poi sono legati ad altri provvedimenti che inevitabilmente caratterizzeranno i nostri confronti nei prossimi mesi. Il PNRR, presidente Gasparri e mi dispiace che questo tema non sia stato colto dal Governo e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ieri in Conferenza dei Capigruppo - non è un piano burocratico che modifichiamo con qualche emendamento per rimetterci a posto la coscienza: è il più grande piano di investimenti, con la chiara finalità della riduzione delle diseguaglianze, che riguarda il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna e tutte quelle aree in ritardo di sviluppo per le quali abbiamo ottenuto quelle risorse. La *governance* del PNRR è stata più volte dibattuta nei due rami del Parlamento e aveva alcune caratteristiche. Per alcune settimane il ministro Fitto ha scaricato sulle caratteristiche dell'impianto generale la colpa di ritardi che in realtà sono ascrivibili solo ed esclusivamente al caos in cui è la maggioranza e, da quel momento in poi, è partita la raffica di dichiarazioni. Ci sono componenti della maggioranza, soprattutto della Lega - il collega Molinari alla Camera che dicono che addirittura potrebbero essere restituite alcune risorse. Altri colleghi di altri partiti della maggioranza dicono che in realtà forse è necessario cancellare alcune finalità, per spostare quelle risorse su altri pilastri del PNRR. Ricordo ai colleghi che i punti fermi del PNRR sono sulla transizione ecologica, sulla transizione digitale, sulla

Ieri sera in Commissione, a testimonianza del fatto che era necessario farlo tutta la settimana e che sarà necessario lavorare ancora la settimana prossima, tutte le risposte che aspettavamo legate al ruolo degli enti locali e delle Regioni non solo non sono arrivate, ma vanno in direzione opposta. Delle due l'una, presidente Gasparri: o la maggioranza ha deciso - e lo chiediamo al Ministro qui presente che quello è un piano burocratico, oppure è evidente che i tempi che ci avete dato e per i quali noi abbiamo contestato il calendario non sono assolutamente adeguati. Aggiungo che noi

noi tutti - sulla necessità di condividere e di impegnare il Senato nell'adottare iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e del senso di appartenenza. Non le sfuggirà, presidente Gasparri, che l'abbiamo presentata per porre un punto fermo su un tema che riguarda tutti noi e la nostra responsabilità, perché eravamo tutti qui il primo giorno della legislatura quando, di fronte alle parole della senatrice a vita Liliana Segre, ci siamo tutti ritrovati. È evidente che, a corrente alternata, autorevoli esponenti della maggioranza e rappresentanti delle istituzioni,

Presidente Gasparri, quella mozione serve a far sì che il Senato si ritrovi intorno a quelle parole. Noi avevamo chiesto di discuterla subito,

le istanze delle autonomie locali sono state di fatto umiliate, come si vedrà nel dibattito pubblico anche fuori dal Senato. È una discussione che a noi sta cuore, presidente Gasparri. Chi rappresenta le istituzioni italiane ha il dovere di farlo sempre e comunque con sobrietà, onore e disciplina, riconoscendosi nella nostra Carta costituzionale, che è il testamento di 100.000 morti caduti nella lotta per le libertà, come ha ricordato Liliana Segre proprio in questa sede nel suo discorso, citando non a caso Piero Calamandrei. Signor Presidente, aver voluto svilire i fatti di via Rasella vuol dire non solo tentare di riscrivere male la nostra storia, ma anche offendere la nostra intera comunità. Ecco perché anche aver parlato genericamente di italiani e non di antifascisti ed ebrei, perché, sì, erano antifascisti ed ebrei...

Quei partigiani erano dalla parte giusta, signor presidente Gasparri. Sono sempre stati dalla parte giusta. *(Applausi)*. Voglio ricordarlo a tutti i nostri colleghi. Se si travisa questo, e a farlo sono i rappresentanti del Governo e delle Istituzioni, non solo si falsifica la storia, ma si rischia anche di non raccontarla bene soprattutto ai ragazzi di oggi. Signor Presidente, le camicie nere non torneranno. Dobbiamo tenere fermi i capisaldi della nostra storia e della nostra Repubblica, perché oggi chiudo con una proposta - il germe del fascismo si nasconde in molte intolleranze che non c'entrano nulla con quegli anni, ma che noi abbiamo il dovere di evitare; esattamente come chi non vuol più punire il reato di tortura, chi non vuole lasciare i minori in carcere, chi vuol dare la colpa di Cutro a chi è morto in mare. Ecco, tutte queste cose sono fascismi e noi tutte queste cose, signor Presidente, abbiamo il dovere di evitare che avvengano quando discuteremo di quella mozione, ricordando cosa a noi tutti? Ricordando che il 25 aprile è la Festa della

come il nostro Paese e la sua storia meritano di essere ricordati. La nostra proposta, presidente Gasparri, è di concedere la prossima settimana di tempo al lavoro che dobbiamo svolgere a partire da giovedì sul decreto PNRR. Oggi abbiamo accettato - mi pare

22 aprile, tra il 20 e il 22 aprile. Chiedo ai Gruppi di condividere la data; ovviamente più colleghi saranno presenti,

Come si può non comprendere che il PNRR potrebbe essere effettivamente per il nostro Paese un'occasione straordinaria di volano addirittura mettere in discussione l'opportunità di utilizzarne le risorse? Seguiamo attoniti i dibattiti che attraversano in queste ore le forze di maggioranza.

Boccia, l'esigenza di avere un momento di approfondimento serio sulla mozione che ieri abbiamo voluto presentare, con le firme di tutti i Capigruppo dell'opposizione. Presidente, voi potete minimizzare quanto volete; potete far finta di non capire quello che l'opposizione in particolare sta cercando di dire in queste ore, ma che pensiamo dovrebbe essere un terreno che interroga tutto il Parlamento, perché riguarda non semplicemente una parte degli italiani, ma tutti gli italiani. italiani. Lo dico anche con riferimento alle dichiarazioni dal mio punto di vista totalmente sbagliate che il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, ha voluto rendere nel corso delle scorse settimane: quando si dicono quelle cose e quando si fanno quelle affermazioni, non si offende soltanto una parte del Paese, ma si offende tutto il Paese, si offendono tutti gli italiani.

quello di seconda carica dello Stato, il discredito che si produce con una dichiarazione sbagliata non è riferibile semplicemente alla persona che lo ha espresso, ma è riferibile all'istituzione che quella rappresenta. È un dettaglio non di secondo piano che penso vada ricordato sempre. In quest'ottica, credo che la discussione che proponiamo a tutto il Parlamento, con la mozione che abbiamo presentato, possa avere tutto il tempo e tutto l'approfondimento che richiede.

credo sia utile separare, altrimenti non rendiamo un buon servizio nemmeno alla possibile intesa che è nostro dovere ricercare. La prima valutazione è relativa ai tempi con i quali si è discusso e affrontato il tema del PNRR e su questo i Capigruppo, anche della minoranza, sanno che il Gruppo del terzo polo polo non ha condiviso questa critica. Non dico che siamo soddisfatti, perché di meglio si può sempre fare, ma abbiamo ritenuto che il percorso in Commissione stia andando avanti e ci porterà, la prossima settimana, all'approvazione dell'atto. C'è poi l'altra questione della calendarizzazione di una mozione delle minoranze, che anche il terzo polo ha firmato e nella quale ci riconosciamo pienamente, rispetto alla necessità di condividere le valutazioni come Senato, nella celebrazione e nel riconoscimento di date fondamentali per il nostro Paese. È del tutto evidente che questa mozione deve essere votata prima del 25 aprile: su questo non ci piove.

della presenza di una persona che, per quella discussione e per tutti noi, ha un valore fondamentale. Quindi, quello che mi permetto di aggiungere alle considerazioni del senatore Boccia quelle date, nella disponibilità della Presidenza, del presidente La Russa e di chi ora presiede l'Assemblea, sulla base anche della possibilità della senatrice Segre di partecipare e di condividere con noi quel momento importante. Questo mi sembra un modo per

le date, come lei sa, possono essere ulteriormente modificate dalla Conferenza dei Capigruppo o da qualsiasi decisione. Non possiamo votare l'auspicio di farlo quando sarà possibile, perché questo disattenderebbe la volontà di discutere la mozione. un auspicio o un impedimento, siamo qui e possiamo sempre ulteriormente modificare. Lo vorrei dire per chiarezza: dobbiamo votare una proposta di calendario.

Signor Presidente, a questo punto, sentite le parole degli esponenti dell'opposizione, facciamo noi una proposta alternativa di calendario, che tenga presente quello che era stato deciso a maggioranza in Conferenza dei Capigruppo. espunge la discussione della mozione nella giornata di mercoledì prossimo, 12 aprile, come era stato stabilito, e si mantiene tutto il resto, con l'impegno

fissare al giorno 20 aprile la discussione della mozione, per avere comunque una data che ne garantisca l'esame prima del 25 aprile. Da oggi fino ad allora, la Conferenza dei Capigruppo e le eventuali intese tra i Gruppi e la Presidenza

«Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure», collegato alla manovra di finanza pubblica. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere

Adolfo ed altri Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese. Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per 1a presentazione dei provvedimenti collegati 21 gennaio, non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che, tuttavia, il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022. Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e delle competenze delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica». Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del del disegno di legge collegato, n. 571, non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

la Commissione finanze e tesoro non è riuscita a completare l'esame del provvedimento, che quindi arriva in Aula senza mandato al relatore. colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Garavaglia, il disegno di legge n. 636, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, del Regolamento. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

di spostare e differire i termini per la discussione di cose importanti. Presidente, non è senza imbarazzo che mi ritrovo nuovamente a intervenire in Aula in questa infinita discussione sui bonus edilizi. Presidente, se ho fatto bene i calcoli, siamo alla ventiquattresima modifica legislativa Presidente, ho una brutta notizia per chi ci sta ascoltando: temo che non sarà l'ultima. Quello che stiamo facendo in questo momento (quello che state facendo) è differire sostanzialmente dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale è possibile completare i lavori ammessi a fruire della detrazione del bonus 110. Sostanzialmente non stiamo dando una risposta definitiva, ma stiamo nuovamente prendendo tempo. Stiamo dando tempo, perché ci siamo resi conto (vi siete resi conto) il blocco della cessione dei crediti ha determinato non solo un problema di liquidità per le imprese e non solo un problema di cassetti fiscali pieni che non si riescono a smaltire, a smaltire, ma anche sostanzialmente, come era prevedibile, il blocco dei lavori. Tanti cantieri aperti, ma in realtà tanti lavori di fatto sospesi.

di maggioranza. E ve l'avevamo già offerta dopo avere sentito in audizione le banche, le imprese e i costruttori. La soluzione che vi avevamo offerto era quella di utilizzare la compensazione degli F24, in cui la banca sostanzialmente non paga solo le proprie tasse all'erario, ma anche le tasse per conto dei propri correntisti, tramite gli F24. Quella era la soluzione - si ricorderanno si ricorderanno i colleghi dell'Aula che questa discussione l'avevamo già fatta a novembre - per non perdere ancora inutilmente altro tempo. Ma non l'avete voluta accogliere. Vi avevamo detto: guardate che, senza quella soluzione, ci ritroveremo tra qualche mese a dover affrontare di nuovo il problema dello sblocco della cessione dei crediti. Eccoci qua, Presidente, siamo di nuovo in questo eterno ripetersi delle cose e siamo ancora qui a offrire tempo, a dare tempo, senza dare una risposta definitiva. Vede, Presidente, io credo che si possano fare delle scelte legittime e che ci siano ovviamente diverse opinioni sul tema del superbonus. Io mi sono già pronunciato e aggiungerò un altro elemento che ovviamente a novembre non potevamo avere, ma che è di tutto interesse: la relazione della Banca d'Italia. Ma il tema che ci siamo posti, cioè quello di risolvere almeno il problema dei crediti fiscali incagliati,

edilizie e coloro che attivano una complessa procedura come quella del bonus della ristrutturazione per il 110. Ci chiedono certezza del diritto, ci chiedono stabilità nel poter fare investimenti. Modificando per l'ennesima volta la normativa - e, ripeto, non sarà l'ultima - non facciamo altro che creare disorientamento negli investitori e questo è un messaggio molto pericoloso, perché non diamo certezza ai rapporti giuridici. Quando

Quando la Banca d'Italia ci dice che ci vogliono quarant'anni per ammortizzare i costi di questa misura significa, signor Presidente, che questo non è stato un buon affare per la società italiana. Quando ci dicono che anche i risultati conseguiti in termini di efficienza energetica e in termini di risparmio di CO2 sono minimali rispetto all'utilizzo delle risorse, tutto questo ci dice che non è stato un buon affare neanche per l'ambiente. dunque di razionalizzare il *bonus* del 110 per cento, l'idea di introdurre una selettività per cui potessero beneficiarne soprattutto coloro che ne avevano più bisogno o gli edifici messi peggio dal punto di vista dell'efficienza energetica o dal punto di vista antisismico era una misura necessaria. Tuttavia, l'idea di bloccare la circolazione dei crediti dall'oggi al domani ha determinato il fatto che abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca, cioè a un problema ne abbiamo aggiunto un altro. Ed è questo il tema che oggi ci troviamo ad affrontare con la proposta che ci viene data. Certamente all'interno della proposta ci sono cose di buon senso, come per esempio la reintroduzione della facoltà di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche: ricordo che questo provvedimento, presentato da me e dalla collega Giusy Versace, proprio la possibilità di detrarre l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è un altro dei *bonus* edilizi che va a scadenza, è stato approvato anche grazie alla maggioranza nella legge di bilancio. In queste cose però, signor Presidente, c'è bisogno di stabilità. In un Paese longevo come il nostro, che sperimenta forme di inaccessibilità, è mai possibile che dobbiamo prorogare di anno in anno misure come le detrazioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche? È mai possibile che dobbiamo introdurre la facoltà di poter utilizzare la cessione del credito, visto che lo stiamo bloccando per gli altri interventi? Signor Presidente, a furia di intervenire su questi *bonus* per 24 volte, non solo se ne va la voce di chi sta intervenendo, ma penso che se ne stia andando anche la voce di moltissimi operatori del settore che sono stanchi di avere continue modifiche normative. Il mio timore è che tra sei mesi ci ritroveremo di nuovo qui.

perché non provate a ragionare sull'unica vera misura che può sbloccare i crediti fiscali incagliati, vale a dire l'utilizzo in compensazione degli F24? Non è una misura a favore del sistema bancario e creditizio, è una misura a favore del sistema Paese. Signor Presidente, colleghi, c'è una ragione per la quale Forza Italia da subito ha posto il tema di una correzione del decreto-legge così come in verità abbiamo fatto a febbraio dell'anno scorso quando il Governo Draghi, dall'oggi al domani, ha limitato le cessioni a una soltanto. La ragione è che lo Stato non può venir meno alla parola data, che lo faccia un Governo o un altro, ed è nostro dovere fare in modo che la fiducia dei cittadini non venga riposta invano. Pertanto si può cambiare idea, si può ritenere non più attuale una normativa, ma si devono salvaguardare i diritti acquisiti e si deve rispettare quel principio europeo dell'affidamento comunemente condiviso, che porta i cittadini a fidarsi del proprio Stato, degli impegni che vengono inseriti da uno Stato nella propria legislazione. Pertanto non potevamo e non possiamo venir meno agli impegni presi. Certo i superbonus hanno generato costi importanti, come sappiamo tutti per averlo verificato; tuttavia non possiamo guardare solo ai costi, dobbiamo considerare anche i benefici, fatti di crescita di PIL e quindi di incrementi degli introiti di imposte e di IVA e di aumenti dell'occupazione. Sono tutte cose delle quali il nostro Paese aveva e ha tuttora estrema necessità. Per queste ragioni si doveva intervenire correggendo una normativa che era diventata ingiustamente penalizzante. Certo rimangono tante criticità

dobbiamo riuscire a fare in modo che le correzioni e i blocchi che ci sono stati non penalizzino i cittadini e non mettano in discussione la parola data, gli impegni presi dal nostro Paese. Sono quindi quindi positive le modifiche apportate alla Camera che, con l'esame in Commissione e poi in Aula, ha aggiunto una disposizione di esclusione dalla responsabilità solidale dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da un intermediario finanziario; la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di utilizzare detti crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, come lo è proroga al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. modo condividiamo la remissione *in bonis* destinata ai contribuenti che non rispettino il termine attualmente fissato al 31 marzo 2023 per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale, relativamente alle spese sostenute nel 2022 e, per le spese sostenute nel 2022, la possibilità per il contribuente di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta 2023. Al tempo stesso il decreto-legge blocca il mercato delle cessioni e degli sconti in fattura a partire dal 17 febbraio 2023, ma salvaguardando i lavori in corso e con importanti esclusioni dal blocco delle cessioni. sono state apportate nella direzione di salvaguardare i contribuenti e il cittadino che si è avventurato su

Per questa ragione Forza Italia sostiene il provvedimento in esame, così come sosterrà eventuali altre modifiche che vadano nella direzione di tutelare l'interesse dei cittadini.

Governo, poiché sono abituata a chiamare le cose con il loro nome, dico subito che oggi siamo chiamati a votare un pessimo decreto. Pessimo per una serie di ragioni; per l'*iter* che lo ha accompagnato, esageratamente veloce, la fiducia, i pareri che non sono arrivati. Un decreto figlio della scarsa visione e della disonestà intellettuale; un decreto che non risolve i problemi e che ha solo lo scopo di attaccare il meccanismo economico della cessione dei crediti di imposta, vero polmone finanziario del superbonus e degli altri *bonus* edilizi. Proviamo per un attimo ad inquadrare lo scenario in cui è nato il meccanismo della cessione dei crediti. Il meccanismo innanzitutto è nato grazie al MoVimento 5 Stelle. Questo è il suo grande difetto, il peccato originale. È nato inoltre in una situazione inedita per il nostro Paese. Ora non lo ricordiamo più, voi non lo ricordate più, lo avete dimenticato presto; eravate quelli che contestavano con facilità ogni provvedimento. Noi invece eravamo quelli che hanno dovuto gestire la pandemia e creare le condizioni per il ritorno alla normalità. Il superbonus nasce in quel contesto, mentre voi stavate a guardare. La quotidianità era stata stravolta, l'economia era ferma, le aziende chiudevano e si preparavano a ridimensionamenti drastici. Un Paese intero era in recessione. Noi, non voi, avevamo la responsabilità di traghettare l'Italia fuori da una situazione improvvisa, assurda ed impensabile. Dovevamo farlo con una misura forte, uno *shock*, e dovevamo farlo agendo su un settore che strutturalmente, per definizione, quando riparte fa ripartire l'intera economia: l'edilizia. Dovevamo ridare battito all'economia italiana; il superbonus, con la cessione dei crediti, è stato il nostro defibrillatore. Ora voi non lo ricordate, non lo volete ricordare, ma le cose sono andate così. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nasce per ridare slancio al settore produttivo mediante un intervento di spesa pubblica che, da un lato, rilanciava il settore edile e, dall'altro, favoriva gli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Anche questo avete dimenticato, perché non avevate responsabilità, non ve non ve le siete mai assunte e potete permettervi l'uso di dimenticare. Fino allo scoppio della pandemia la vera emergenza si chiamava, e purtroppo si chiama ancora, cambiamento climatico e prima che il presidente Giuseppe Conte imponesse all'agenda europea il Next generation EU, in cima all'agenda c'era il Green deal. Da qui nasce il superbonus, con la cessione dei crediti; una misura che permetteva di rilanciare un settore economico e perseguire gli obiettivi climatici, pur in una fase di recessione economica. Una misura coraggiosa e geniale, proprio così, che ha generato un impatto potente sul tessuto economico e occupazionale del nostro Paese. Una misura a cui avevano accesso tutte le fasce di reddito, anche le più fragili e con minore capacità di spesa. È questo che un Governo deve e dovrebbe fare quando il suo popolo vive un periodo di profonda crisi e disperazione, quella vera. *(Applausi)*. È di questo che stiamo parlando. Tutto dimenticato. Bravi. Con la cessione dei crediti il Paese è ripartito con alla base l'intenzione e la volontà di non lasciare nessuno indietro. Tutto questo accadeva mentre voi stavate a guardare. Questo nella fase uno. Nella fase due, quella che è diventata maggioranza ha iniziato a raccontare falsità, ha iniziato a lanciare accuse e critiche, tutte infondate, sulla cessione dei crediti e del superbonus. Ricordo, Presidente, visto che qui si continua a fingere di dimenticare, che lo strumento della cessione dei crediti ha generato un milione di di posti di lavoro e un aumento del PIL del 7 per cento nel 2021 e del 3,7 per cento nel 2022; qualcosa di eccezionale, di cui tutti dovremmo essere orgogliosi. La misura andava difesa, protetta e accompagnata con cura. la scelta è stata quella di frenare la crescita, la ripresa di un settore al quale era stato dato finalmente l'ossigeno che necessitava. È stato deciso di strappare via improvvisamente la spina per farlo morire. Questo Governo è palesemente in preda alla smania di cancellare le misure di successo. Come se cancellare, dimenticare, sminuire e delegittimare il lavoro fatto bastasse a far apparire sufficiente il vostro scarso lavoro di questi mesi, condito di propaganda ideologica. Prima di evidenziare l'impatto, a mio avviso, ripeto e insisto, disastroso di questo provvedimento, voglio ripercorrere l'evoluzione del meccanismo della cessione dei crediti. Nell'ordine, l'articolo 121 del decreto-legge n. 34, del 2020, che questo provvedimento stravolge, è stato modificato ben diciotto volte; due volte nel 2020, durante il Governo Conte II, volte durante il Governo Draghi e ben tre volte dall'insediamento dell'attuale Governo. Addirittura le ultime due modifiche intervengono a distanza di un mese l'una dall'altra. E meno male che non volevate disturbare. Come pensate di attrarre investimenti o di fornire garanzie e certezze normative alle imprese in questo modo? Non c'è immedesimazione, non c'è la volontà di fare proprie le difficoltà di imprese e famiglie, ma solo quella di soddisfare una schizofrenica bulimia normativa che imprese e famiglie dovrebbero inseguire, ma non è possibile farlo. Per quanto riguarda il decreto, la nostra contrarietà non è data dal fatto che la cessione dei crediti sia una nostra misura e quindi ci siamo rimasti male. No, questo è il vostro stile, non è il nostro. Noi non anteponiamo bandierine agli interessi di imprese e famiglie. Presidente, la nostra contrarietà è rivolta alla diciottesima modifica, perché oltre a generare ancora più confusione distrugge una delle poche politiche di spesa che ha generato lavoro, reddito ed efficientamento energetico privilegiando l'*austerity.* Presidente, mi perdoni se insisto, ma vi siete presentati alle urne come l'alternativa all'austerità, salvo poi rivelarvi la brutta copia di Draghi. In tutto questo, a pagare il prezzo di è stato certificato: la cessione dei crediti altro non è che il meccanismo tramite cui rendere fruibile a tutti, anche alle classi sociali economicamente più fragili, i meccanismi di efficientamento energetico energetico degli edifici e questo non lo dice Sabrina Licheri, non lo dice il MoVimento 5 Stelle, ma lo dicono sia l'Ufficio parlamentare di bilancio, sia Bankitalia: la cessione dei crediti fiscali era un meccanismo in grado di venire incontro ai più deboli. *(Applausi)*. lo ribadisco - è stato il defibrillatore, il farmaco salvavita, ma voi siete come quelli che, scampato il pericolo, contestano la cura e ne sminuiscono gli effetti. Quando però non potevate permettervi di contestare la cura perché avreste perso il voto degli italiani, che misurano le politiche in base alle vere ricadute che queste provocano sulla quotidianità, quando non potevate permettervi di contestare il superbonus non per onestà intellettuale, ma per mero calcolo elettorale, era divertente girare i video dove venivano condannati i quindici interventi di modifica della normativa ad opera del Governo Draghi. Per non parlare poi di quelli nei quali si chiedeva lo sblocco dei crediti incagliati. Anche questo è dimenticato? Era divertente, ma soprattutto era facile fare opposizione. Sempre quando non potevate permettervi di contestare il superbonus, il programma di Forza Italia proponeva il rinnovamento del patrimonio edilizio. La stessa Forza Italia che alla Camera aveva presentato una mozione di otto pagine, con otto impegni al Governo per tutelare il superbonus e la cessione dei crediti. Poi, il giorno dopo le elezioni regionali, dando uno schiaffo al vostro elettorato, in maniera subdola presentate un decreto sulla cessione dei crediti fiscali che non presenta uno straccio di cessione dei crediti fiscali. Un problema su tutti doveva essere risolto, quello dell'incaglio dei crediti d'imposta impantanati nei cassetti fiscali di decine di migliaia di aziende

di categoria come ANCE e CNA. Non solo, ma avete gettato le imprese in una situazione di non ritorno per un vostro mero giochetto politico, ma dopo le avete anche accusate di parzialità. Peggio ancora, giustificate l'eliminazione della cessione dei crediti con il discorso delle frodi, come dire che vanno eliminate le pensioni di invalidità per eliminare i finti ciechi beccati alla guida di autobus. Quando una politica pubblica genera o può generare comportamenti fraudolenti si interviene con meccanismi che li contrastino e li blocchino, non si blocca lo strumento. Il superbonus rappresenta soltanto il 5 per cento sul totale delle frodi commesse in materia di cessioni dei crediti. Questo vuol dire che è possibile prevedere un meccanismo di cessione dei crediti che non si presti E anche questo non lo dico io, lo ha detto l'Eurostat. Da ultimo, oltre al danno la beffa: mi riferisco alla direttiva casa *green*, che prevede la riqualificazione di circa 1,8 milioni di abitazioni entro il 2030 e il 2033. La direttiva *green*, che vi piaccia o no, prima o poi dobbiamo affrontarla e rispettarla e la strategia non può certo non può certo essere quella di chiedere proroghe su proroghe. Prima o poi dovremo affrontarla e agire e per farlo dobbiamo garantire che nessun cittadino venga lasciato indietro. Lo dobbiamo Lo dobbiamo fare attraverso lo strumento della cessione dei crediti, e l'unico meccanismo che permette di convertire il patrimonio italiano in un'ottica di efficientamento energetico lo avete buttato via. State deliberatamente soffocando il necessario percorso verso la rigenerazione e la sostenibilità ambientale delle nostre città, per non parlare delle periferie e delle aree più interne, più interne, o dei 170.000 posti di lavoro a rischio. Meno male che non volevate disturbare chi aveva voglia di lavorare e soprattutto meno male che eravate pronti. Auguri a tutti noi e non solo di buona Pasqua. *(Applausi)*.

Signor Presidente, ci troviamo a discutere un decreto-legge che è sicuramente importante, visto quello che è successo negli ultimi mesi. Come abbiamo detto sin dal principio, oggetto era una misura che per certi versi poteva essere d'aiuto, ma doveva essere strutturata in maniera ben diversa. Così come era stata strutturata, era evidente che avrebbe prodotto degli incentivi in maniera perversa, una distorsione del mercato e una distorsione della libera concorrenza dei prezzi e che avrebbe prodotto purtroppo una circolazione illimitata dei crediti, che

siamo arrivati a questa situazione assai complicata. Abbiamo visto che sono già stati accertati

Detto questo, è stato appunto opportuno intervenire, con un provvedimento sicuramente non semplice, ma che pone dei punti ben fermi. Ne cito alcuni: l'articolo 01 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento fino al 30 settembre 2023,

solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei concessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, ad utilizzare questi crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. Ferma poi restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari alla violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito d'imposta e siano in possesso di specifica documentazione, tra cui una attestazione riguardante il rispetto delle norme anti-riciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni. Il decreto inoltre chiarisce che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce da solo causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario e l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave grava sull'ente impositore. quindi tutta una serie di disposizioni che proseguono con l'articolo 2, che stabilisce, a partire dal 17 febbraio di quest'anno, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta

e quelli danneggiati da eventi meteorologici verificatisi, ad esempio, nella Regione Marche. Quindi il decreto-legge al nostro esame è assai complesso. Contiene tutta una serie di norme di interpretazione autentica che chiariscono che per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo e che anche l'indicazione, ad esempio, delle spese sostenute per il rilascio del certificato di conformità costituisce una mera facoltà e non un obbligo. Ci sono poi alcune disposizioni in favore del contribuente che può avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis* e tutta un'altra serie di disposizioni che mirano a fare chiarezza in quella che era diventata una vera e propria giungla. Il Governo si è trovato in una situazione assai difficile e questo è ben dimostrato - lo ripeto dalle truffe già accertate e dai 19 miliardi di crediti incagliati. È evidente che bisognava mettere mano a questa nuova normativa, purtroppo per l'ennesima volta. Non abbiamo ovviamente la pretesa di avere risolto tutti i problemi tramite questo provvedimento, ma riteniamo di aver preso la la strada giusta *in primis* per mettere in sicurezza il bilancio pubblico e poi anche per proteggere quelle imprese e quelle famiglie che si sono avvalse di una legge dello Stato e che non devono assolutamente essere penalizzate. Ritengo quindi che quello al nostro esame fosse un decreto urgente. Ritengo che queste misure vadano tutte nella direzione di salvaguardare imprese, famiglie e conti pubblici e quindi il nostro il nostro Gruppo darà il proprio appoggio convinto all'approvazione del decreto-legge al nostro esame che finalmente mette mano e risolve una buona parte dei problemi che si sono venuti a creare nel corso di questi ultimi mesi.

dall'inizio di questa legislatura. Ho già avuto l'opportunità di dire che la toppa che avevamo messo apriva una voragine e siamo di fronte a questo,

la responsabilità - sottolineo: la responsabilità - di aver portato questa situazione alla paralisi, perché il giorno stesso che si è insediato e abbiamo svolto una discussione sulla NADEF, ha attaccato e ha deciso che il superbonus andava abolito.

che era necessario ed è necessario. Questa è la cosa che vorrei sottolineare: è necessario affrontare il problema di come noi rispondiamo all'Europa. Certo voi siete andati in Europa a mostrare i muscoli, dicendo che il 2035 o il 2050

al patrimonio urbanistico del nostro Paese. Se vogliamo mettere a disposizione delle giovani generazioni e degli anziani alloggi sufficientemente confortanti, dove sia

non si lavora e ci sono crediti incagliati, ma anche la difficoltà di imbarcarsi in una situazione in cui non si sa se si può iniziare e come si può finire, perché si continuano a cambiare le norme. Invece, bisogna dare norme certe, per evitare le speculazioni. La soluzione ve l'avevamo proposta: erano gli F24.

scaricare nella propria dichiarazione dei redditi. Quindi, siamo di fronte al fatto che quelli che hanno manifestato la settimana scorsa, avendo ragione,

salta ovviamente la decisione presa e questo crea ritardi enormi. Pensate all'impresa che ha i ponteggi in affitto fermi

ed è per questo che io credo che anche la proposta che avete fatto, che tenta almeno alcune correzioni, da un punto di vista tecnico non risolve niente. Quindi, vi invito a rivedere e a discutere in modo molto in modo molto meno ideologico. Voi avete assunto questo tema in modo ideologico. D'altronde, è vero: siete un Governo politico; ideologicamente siete contro il progresso ed è per questo che avete affrontato con questo piglio il tema del superbonus.

senatrici e senatori, Governo, durante la campagna elettorale per le passate elezioni politiche, nel tripudio di retorica che ha contraddistinto la sua strategia comunicativa, l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiarava pieno sostegno e sicuro aiuto, in caso di vittoria, a tutti coloro che in questi anni hanno investito sui bonus edilizi, che hanno formato le proprie maestranze, che hanno innovato i propri studi professionali per stare al passo con la normativa. Vinte le elezioni - e dunque potremmo dire, con un linguaggio popolare, "passata la festa" - tutte le promesse sono state archiviate; anzi, molto peggio, sono state stravolte. Per dare la misura di queste mie affermazioni, potrei qui ricordare anzitutto le dichiarazioni del ministro dell'economia Giorgetti e della stessa presidente Meloni, che, a favore delle telecamere, dissero che la cessione dei crediti fiscali non era un diritto. Tale dichiarazione, da una parte, gettò nello scompiglio un intero comparto produttivo, ma, allo stesso tempo, chiarì in modo inequivoco e definitivo l'intendimento demolitorio del Governo in materia di crediti fiscali e di bonus edilizi. Poi dalle dichiarazioni si è passati ai fatti e con il primo decreto-legge aiuti del Governo Meloni si è introdotta la tagliola del 25 novembre. Dovremmo ricordare tutti come la decisione del *décalage* e di quella data-mannaia generò una corsa una corsa verso gli uffici tecnici comunali di tutto il Paese, per presentare la documentazione tecnica valevole per l'ottenimento dei benefici di legge. Furono giorni di totale confusione e - lo ricordano bene imprese e professionisti - nottate di lavoro per sapere di quale morte sarebbero deceduti progetti e speranze delle famiglie. La protesta montò in modo forte e fu sempre più chiaro a tutti che il Governo della destra si assumeva la responsabilità di rompere il patto di lealtà con i cittadini contribuenti e con la loro fiducia riposta nelle istituzioni. Mai avremmo dovuto dare, dalle Aule parlamentari e dalle stanze di Governo, la sensazione che si possono cambiare le regole in corsa, facendosi beffa dei sacrifici di chi sulla propria casa stabilisce le fondamenta della crescita della propria famiglia. Ma il piano inclinato non si è interrotto e nelle settimane successive, andando verso la discussione della manovra di bilancio e poi del decreto-legge milleproroghe, la musica non è cambiata. Abbiamo assistito solo a improvvisazioni, a salti nel vuoto normativo e a piroette di chi, da una parte, introduce norme molto penalizzanti e dall'altra, nel giro di poche ore, torna indietro, modifica e rettifica. È esattamente questo il *modus operandi* con il quale si è buttato nella mischia, come un fulmine a ciel sereno, il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il cosiddetto decreto crediti. Ricordo benissimo - e dovrebbero ricordarlo anche i colleghi e le colleghe di maggioranza - che, nelle ore subito precedenti il Consiglio dei ministri chiamato a deliberare, non appena iniziarono a circolare le bozze del testo normativo, le reazioni delle associazioni di categoria, delle imprese, degli artigiani, degli esodati del superbonus e delle professioni tecniche presero letteralmente d'assalto tutti noi rappresentanti delle istituzioni, nazionali e locali. Nessuno poteva e voleva credere ai propri occhi, ma di fatto è accaduto questo: per mesi si è atteso un provvedimento che risolvesse il problema del blocco dei crediti, il quale inchioda nei cassetti fiscali decine di miliardi di euro, bloccando a sua volta un intero comparto e togliendo il sonno a tante e tanti, ma, contrariamente a quest'attesa, si stava approvando un decreto che più opportunamente potremmo chiamare blocca crediti o blocca edilizia. Con un colpo di spugna avete eliminato sconto in fattura e cessione del credito e non avete introdotto alcuna misura vera per l'alleggerimento dei pacchetti dei cassetti fiscali. Avete fatto persino di più: anche per i territori del cratere sismico 2009-2016, dopo paginate di promesse, avete eliminato la facoltà di utilizzo della cessione dello sconto. Dal momento della deliberazione del Consiglio dei ministri in poi, abbiamo assistito al solito psicodramma già visto già visto per tutti gli altri provvedimenti del Governo: annunci di interlocuzioni, promesse di modifica, riunioni interminabili e divisioni nella maggioranza, mentre il Paese, fuori dai luoghi della decisione, osservava preoccupato e ansioso. Vi siete presi un mese e mezzo di tempo, lasciando tutti sospesi, per fare macchine indietro. È così che su nostra sollecitazione avete reintrodotto lo sconto in fattura, la cessione per gli immobili dell'ex per le cooperative e per le opere riguardanti le barriere architettoniche. È servita una battaglia parlamentare di territorio per farvi capire che sui crateri sismici questo decreto sarebbe stata una sciagura e stupisce che non ne fossero avveduti i senatori e le senatrice provenienti da quella terra. Solo così avete reintrodotto anche per questa fattispecie gli strumenti normativi originari. Tuttavia, l'ho già detto e lo ripeto, il miglior modo di risolvere i problemi in genere è non crearli. punto se si può assistere ad articoli di stampa di giubilo per aver reintrodotto cessione del credito e sconto in fattura nel cratere sismico. Non sarebbe bastato lasciare le norme com'erano, senza modificare per poi rimodificare, con almeno il buongusto di non gioire per aver fatto un danno a cui solo in parte si è riparato? Osserviamo, inoltre, che il cosiddetto decreto blocca crediti è l'ennesimo esempio di un'offesa al parlamentarismo da parte della maggioranza, che ormai costringe le nostre Assemblee a discutere solo di decreti-legge con tempi serratissimi e senza la profondità che una tematica come questa, che sta mettendo a rischio non solo la tenuta economica, ma anche sociale del Paese, avrebbe meritato. Non possiamo che essere contrari a questo provvedimento, non possiamo che essere speranzosi, sebbene fiaccati nelle nostre speranze dal vostro modo di agire, perché tante imprese, tante famiglie e tanti professionisti vedano presto una soluzione definitiva alle loro angosce. Vorrei concludere, signora Presidente, richiamando un punto politico che ritengo essenziale e centrale, che riguarda la dignità della funzione parlamentare. È evidente che siamo ormai in un regime di doppio monocameralismo, per cui questa nobile Assemblea, che dovrebbe rappresentare il popolo, è oggi poco più che un dopolavoro parolaio. Noi esprimiamo infatti opinioni, ma la discussione per chi è fuori da quest'Aula è già finita alla Camera dei deputati. Fuori da qui, per essere sinceri e anche consapevoli, nessuno aspetta la nostra discussione. Lavoratrici, lavoratori e imprese hanno solo capito sostanzialmente tre cose. rimane l'incertezza sui crediti incagliati: dopo sei mesi, dopo che il problema si era posto già con il precedente Governo,

alcuna visione per il futuro sull'efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Come ha detto la senatrice Licheri, prima o poi dovremo discutere, anche grazie alla direttiva sulle case *green*, su cosa l'Italia vuole fare rispetto all'innovazione del proprio patrimonio edilizio e all'efficientamento energetico, che non solo è contrasto ai cambiamenti climatici, non solo è diminuzione del costo delle bollette energetiche direttamente per le famiglie, non solo è generazione distribuita di energia, ma è anche creazione di lavoro buono e nuovo.

e allora, però, dovevamo fare di tutto per ottenere tutte le risorse del PNRR - oppure, se non abbiamo bisogno di quelle risorse, evidentemente non abbiamo un problema di bilancio. Alla fine di questa nostra attività parlamentare con l'orgoglio collettivo di esserci occupati di grandi emergenze sociali come quella dei *rave party* e non di queste che evidentemente sono quisquiglie.

Il provvedimento arriva in Senato a poche ore dalla celebrazione della ricorrenza del sisma dell'Aquila: del 6 aprile ha infatti segnato la storia della città di L'Aquila e di tutto l'Abruzzo. Queste sono le ore dedicate al doloroso ricordo delle 309 vittime e di quella devastazione che ha colpito il nostro capoluogo di Regione e le aree circostanti, una catastrofe le cui immagini restano impresse negli occhi di noi abruzzesi e non solo. Significativa è in queste ore la presenza a L'Aquila del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e di altri rappresentanti istituzionali del Governo. È un segnale di vicinanza importante a una terra che ha dovuto e ha saputo rialzarsi e che ancora oggi fa i conti col tema della ricostruzione. Desidero ricordare il terremoto dell'Aquila perché più volte, quando si è parlato del superbonus in Commissione, ma anche in quest'Aula, si è fatto riferimento alla prevenzione. Dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte a una fragilità diffusa: abbiamo la fortuna di essere nati in una terra meravigliosa come l'Italia, che è bella, ma altrettanto fragile, quindi ci troviamo di fronte a una fragilità diffusa

di non disperdere le poche risorse che ci sono e, se c'è un aspetto che non ho mai condiviso del superbonus e di chi lo ha concepito, è l'aver fatto credere che chiunque potesse ristrutturare gratuitamente la propria abitazione, con una sorta di finanziamento a pioggia, senza introdurre alcun criterio di priorità, che nulla ha a che fare con la prevenzione. *(Applausi)*. Si è cercato di far credere agli italiani l'utopia che nessuno pagava, tutti potevano ristrutturare la propria abitazione e che tutti ci guadagnavano, anche lo Stato. Si che è costata alle casse dello Stato 120 miliardi (per capirci, quasi quattro manovre finanziarie), che ha fatto lievitare i prezzi alle stelle e che ha portato a truffe

imprese e aziende, altro che rilancio economico. Il mio pensiero va a tutte le imprese che hanno

che loro hanno creato e che il Governo Meloni ha ereditato. Questo va detto in maniera chiara, diretta e sincera agli italiani.

oltre a tutte le interpretazioni e le circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate che hanno creato un caos normativo che ha spinto molti cittadini, molti professionisti e molte imprese a non credere mai nel superbonus. Bisognava intervenire? Sì, certo. Bisognava intervenire per cercare di cogliere obiettivi molto importanti; innanzitutto, quello di cercare di salvaguardare i conti dello Stato, a seguito anche del nuovo regolamento di contabilità pubblica di Eurostat, nel quale i crediti d'imposta venivano visti immediatamente immediatamente come spesa e quindi come disavanzo. Bisognava cercare di sbloccare i crediti incagliati.

La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono stati bloccati dal Governo Meloni, ma lo erano già da tempo: nessuno era più disposto ad acquistare i crediti. Questa è la verità. Perché si è deciso allora di lavorare su questo provvedimento? Innanzitutto, non si poteva chiedere al Governo di sbloccare crediti incagliati e contestualmente permettere di crearne altri.

dicevano una cosa estremamente chiara, ossia chiedevano di aiutare a risolvere il problema dei crediti incagliati. Questa misura è presente all'interno del provvedimento, chiarendo le responsabilità di chi acquista i crediti, con l'utilizzo decennale dei crediti d'imposta per le banche e le imprese, la possibilità di trasformare i buoni poliennali del tesoro quali crediti che sono rimasti a fine anno nelle pance di banche ed istituti di credito e la costituzione di una piattaforma per cercare di far incontrare la disponibilità dei crediti con la loro richiesta. Queste prime, sagge iniziative del Governo hanno condotto a comunicati stampa che vanno nel senso sperato: si stanno finalmente sbloccando i crediti incagliati. È un successo che va riconosciuto

un uso non oculato delle risorse, quindi all'interno di questo decreto, grazie anche al lavoro svolto all'interno della Commissione della Camera, si è cercato di dare risposte puntuali a determinate realtà che hanno l'esigenza di riuscire a risolvere alcuni problemi. Mi riferisco ad esempio alle zone del colpite dal sisma e dalle

Ci troviamo di fronte a un decreto-legge nel quale il Governo Meloni si assume la responsabilità di assume la responsabilità di trovare soluzioni a una situazione di caos normativo che le opposizioni hanno creato e che noi intendiamo affrontare con determinazione.

difficili e drastiche, ma arriva il momento di farlo con assoluto e totale senso di responsabilità. Dopo due anni di politica dei *bonus*, con il meccanismo della cessione del credito, è doveroso tirare le somme. La fotografia fatta dagli istituti indipendenti, come l'ufficio parlamentare di bilancio, l'Agenzia delle entrate e la Banca d'Italia, è impietosa: 110 miliardi di crediti edilizi generati in appena due anni, 9 miliardi di truffe accertate un mancato gettito per le casse dello Stato che per i prossimi anni sarà stimato in 8-10 miliardi in meno per ogni annualità. Sul superbonus c'è una sostanziale unanimità nella consapevolezza che la gestione degli incentivi edilizi negli ultimi anni ha provocato una serie di criticità molto importanti. Efficientare, ristrutturare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio è senza dubbio un obiettivo da perseguire. In Italia insistono 12 milioni di immobili, la maggior parte dei quali è stata realizzata prima degli anni Ottanta. Il lavoro da fare è tantissimo, ma dobbiamo prendere consapevolezza che per centrare l'obiettivo occorrono politiche e misure serie, che diano certezza agli operatori e alle famiglie senza esporli a rischi generati da una propaganda politica che spesso è stata a dir poco vergognosa, perché l'essere andati nelle piazze a raccontare alla gente che poteva ristrutturare casa gratuitamente ha reso evidente che, più che perseguire l'obiettivo, si è cercato il facile consenso, illudendola. È questo il peccato originale per cui oggi ci troviamo con la cifra mostruosa di 19 miliardi di crediti incagliati, che pesano come un macigno sulle imprese e sui conti pubblici. Sul principio di equità sociale dobbiamo riscontrare che a beneficiare di più di questi soldi pubblici sono stati quelli che forse ne avevano meno bisogno: proprio il 10 per cento dei contribuenti più ricchi ha potuto fruire della metà dei crediti che sono stati generati. A beneficiare direttamente del 50 per cento degli investimenti sono stati i più benestanti d'Italia. Così, grazie alla politica del «gratuitamente», i ricchi hanno potuto ristrutturarsi le seconde, le terze e le quarte case, al mare o in montagna, con i soldi di tutti i cittadini, anche quelli che non sono proprietari di case. *(Applausi)*. Un intervento così iniquo a favore dei ceti più agiati non si era mai visto. È vero che bisognava far ripartire l'economia ed è vero che ci trovavamo in un periodo gravissimo, quello della pandemia, ed era necessario fare qualcosa per rilanciare per rilanciare le imprese sul nostro territorio, ma si sarebbero dovuti mettere quantomeno dei parametri per facilitare le fasce più deboli e non quelle più abbienti. Gli interventi a favore dell'edilizia residenziale pubblica invece sono stati marginali, quando forse occorreva partire proprio da lì. Sulla produttività dell'investimento, ovvero sui vantaggi che questo tipo di intervento si era proposto di generare, dobbiamo dire le cose come stanno. Se l'obiettivo era quello di abbattere il consumo energetico, i risultati sono stati miseri. Come ha certificato la CGIA di Mestre, a fronte di una spesa di 72 miliardi di euro, è stato riqualificato appena il 3 per cento del patrimonio immobiliare italiano.

Qual è il beneficio reale del risparmio energetico che avremo sul sistema? Praticamente nulla: tanta spesa per nessuna resa. Da qualsiasi lato la si guardi, questa misura assume le sembianze di un macroscopico fallimento, un disastro precedentemente generato dal Governo giallorosso. Gli interventi Gli interventi per gli IACP, per le zone colpite da sisma e alluvioni, le proroghe e tutte le altre norme introdotte contribuiscono ad alimentare quella fiducia che negli ultimi tempi si era ridotta ai minimi termini. Il problema non è di facile soluzione, assolutamente, ma siamo convinti che il Governo saprà dare presto risposta a tutte le famiglie e le imprese che oggi scontano sulla propria pelle una politica dissennata,

oserei dire, un po' parafrasando, grosso come una casa - e una criticità proprio sul terreno dell'incapienza. Il dato è che il decreto-legge

Per quanto riguarda il merito, si è detto che abbiamo risolto. Posso dire che spero che questo provvedimento risolva il

si indicano i crediti e c'è qualcuno che li compra. Ma chi lo fa? Noi abbiamo proposto chi doveva farlo. Avevamo parlato degli F24 oppure di una società pubblica che intervenisse su questo

alla criminalità organizzata, perché in una situazione simile, prima di fallire, si tentano tutte le strade e il rischio è molto alto.

sto parlando di soldi, di risparmi, del fatto che il cittadino investe in questo. Anche qui, però, mi dovete spiegare come poter davvero rilanciare

affinché le persone abbiano fiducia che quello che stanno facendo produce un loro interesse, perché c'è un contenimento energetico, perché la loro casa è più agibile, perché in sostanza c'è una rivalutazione del loro patrimonio. Anzi, questa operazione dovrebbe farla lo Stato, a partire dal suo patrimonio sua messa in sicurezza. Noi siamo un territorio ad alto rischio sismico e tutte le volte che arriva una scossa tremiamo tutti e temiamo che possa succedere qualcosa di più grave. prevenire più che curare. Se vogliamo prevenire, però, bisogna fare un intervento programmatorio. Bisognerebbe pianificare, ma qualcuno potrebbe sostenere che è una parola comunista e quindi non si può dire.

l'idea che in questo Paese, con la spesa pubblica, si possa sostenere e affrontare qualsiasi situazione; l'idea che lo Stato possa pagare le migliorie alla casa, magari pagandole ai cittadini più ricchi, e l'idea che lo Stato possa pagare i cittadini per non lavorare. Perfetto: tutto torna. Queste due teorie hanno contrassegnato le proposte politiche di una forza che si era alimentata di demagogia e che, nel momento di calo, ha in qualche modo rigenerato una quota parte della propria fortuna attraverso questi due interventi. due interventi. Un filo rosso lega questi temi: l'idea di una irresponsabilità verso il sistema Paese, l'idea di un assistenzialismo che ha portato fino all'esasperazione, l'idea di un principio sbagliato di spesa pubblica. Si dice che, però, ha rimesso in piedi l'economia nel campo dell'edilizia. Io penso che rimettere in moto una quota parte di economia, generando quella spesa pubblica e con una misura *una tantum*, sia un pannicello caldo, che ha in sé delle storture. A rimettere in moto l'economia del Paese - lo dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che hanno ideato questa strategia - sono l'alta velocità, le strade, i ponti, i porti, gli aeroporti,

Noi abbiamo da contrastare innanzitutto un'idea di Stato che punta su un eccesso di ruolo nel campo economico e che immagina il tema dei sussidi come un aumento del perimetro del I dati parlano chiaro, non c'è bisogno di inventarseli: il superbonus ha triplicato il costo dell'efficientamento; ha aumentato il prezzo per le ristrutturazioni, perché avere eliminato la concorrenza sul prezzo è stato un elemento di negatività. È l'idea stessa del superbonus 110 che probabilmente ha comportato questo tipo di scenario.

è relativo al superbonus. Quanto aumenta il costo delle detrazioni che abbiamo ingenerato con questo tipo di meccanismo? Circa 70 miliardi. 70 miliardi. È crescita del debito pubblico ed è un qualcosa che poteva essere utilizzato nel nostro Paese con più positività nel campo della sanità, dell'istruzione, della riduzione del costo del lavoro. Penso che qui stia la differenza tra una visione assistenzialista che blocca lo sviluppo del Paese, e che lascia i problemi alle generazioni successive, e i riformisti dei quali mi onoro di far parte. Detto ciò, collega Sigismondi,

senatore Sigismondi, e dovete fare qualcosa. Aver detto in campagna elettorale che questa misura dovesse essere cambiata non elimina due elementi. Il primo è di verità storica: dentro la vostra compagine, la destra, ci sono forze politiche che queste misure comunque le hanno votate. Questo è il primo punto di chiarezza da spiegare ai cittadini. Il secondo elemento:

il ruolo di forza di Governo non elimina la necessità di modificare questo intervento *(Applausi)*, salvaguardando le persone che hanno messo in moto quegli interventi sulla base di norme dello Stato.

che si candida a governare il Paese e che oggi lo sta governando ha il dovere non di dire che bisognava fare qualcosa - come ha detto il senatore - ma di dire cosa bisogna fare. Arrivo al

perché non risolve il problema dei crediti incagliati. Avevamo avanzato una proposta, ossia l'utilizzo del modello F24, oppure l'idea che attraverso garanzie SACE ci possa essere un intervento delle banche più convincente: delle due l'una. Ma certamente non è una risposta dire che si utilizzerà probabilmente la piattaforma Enel X. A tale proposito avrei delle domande da fare sui tempi, modi di attivazione e sulla quantificazione. Sono questioni che dentro questo provvedimento non trovano la chiarezza necessaria, lasciando nell'indeterminatezza cittadini, imprese e famiglie che avranno pure lavorato sulla base di una norma che non è convincente, ma che hanno agito sulla base di una regola. Per quanto

se da un lato il terzo polo condivide una critica pesante a questo tipo di incentivi dati a pioggia, che addirittura ha il paradosso di rimettere a sistema le case dei ricchi pagate dai poveri, cioè Robin Hood al contrario; dall'altro lato, io non me la sento di votare certamente la fiducia, ma nemmeno il provvedimento, perché lascia quelle famiglie, quei cittadini e quelle imprese completamente allo sbando. Questa è, in fondo, la prima dimostrazione che avevate a disposizione per farci capire che qualità e che tipologia

cominciano a stare a zero. E ve lo dice la rappresentante di un Gruppo che non ha utilizzato la demagogia nel rapporto con la maggioranza. se sul PNRR, che è una misura strutturale differente da quello di cui stiamo parlando oggi, e quindi pienamente in linea con quello che io penso sia buono, il vostro lavoro di cambiamento, anziché il primo giorno in cui vi siete insediati, è intervenuto dopo sei mesi, non ne hanno colpa il terzo polo e neanche la minoranza, che fa l'opposizione. La responsabilità è di chi ha probabilmente perso molti mesi in demagogia

che, se c'è la volontà di mettere mano agli errori commessi nel passato, troverete sempre da questa parte dell'opposizione un atteggiamento corretto e propositivo. Se invece la vostra idea di Governo e di continuità amministrativa è lasciare nel caos cittadini, famiglie e imprese, troverete da questa parte dell'opposizione una critica assolutamente netta perché a pagare le spese della vostra incapacità di risolvere i problemi non siano i cittadini, magari i più fragili, magari quelli che hanno la necessità di essere aiutati. Così come diremo anche la prossima settimana, noi continuiamo a pensare che la risoluzione che la risoluzione ai problemi del nostro Paese non passi attraverso i sussidi, non passi attraverso i bonus, non passi attraverso gli interventi a pioggia, ma passi attraverso la capacità di progettare un Paese in modo serio. *(Applausi)*. Lavorate su Industria 4.0, rimettete in piedi la struttura tecnica di missione Italia Sicura, lavorate per contrastare il dissesto idrogeologico: questi sono interventi che aiutano la sicurezza e generano anche una capacità positiva nella nostra economia. E poi, togliete le risorse pubbliche che in questo momento volete utilizzare per rifare gli stadi, perché francamente di questa vostra ossessione per aiutare le squadre di calcio ne abbiamo le tasche piene. *(Applausi)*. Noi vorremmo che le risorse dei cittadini venissero utilizzate per le cose utili al Paese. Ripeto: siete partiti da una critica giusta e siete finiti per avere invece, da parte nostra, una valutazione negativa su quello che state facendo. Non so se è per miopia politica, non so se è per incapacità, ma dopo sei mesi cominciano a preoccuparmi la vostra visione corta del futuro e la vostra incapacità di offrire soluzioni al Paese.

quando venne pubblicato il decreto oggi in discussione, Forza Italia chiese con forza di poterne discutere approfonditamente alla Camera e così è stato. Sono stati tanti gli emendamenti accolti che hanno arricchito e migliorato il testo. Il problema principale che il decreto affronta è lo sblocco dei crediti incagliati che - secondo le ultime stime - ammontano Più volte in quest'Aula abbiamo lanciato il grido d'allarme, temendo che i crediti incagliati avessero portato a migliaia di fallimenti di imprese e alla conseguente drammatica perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Ringrazio il Governo per averci ascoltato. Sfatando anche la narrazione della sinistra, che vuole il centrodestra diviso e litigioso, semplicemente abbiamo posto un problema che andava risolto e il Governo e la maggioranza in Parlamento stanno implementando le strategie per risolverlo. C'era grande difficoltà nel settore bancario rispetto alla responsabilità solidale cui erano chiamate le banche: oggi questo problema viene risolto, prevedendo la circoscrizione del perimetro della responsabilità solidale, qualora siano presentati documenti comprovanti l'effettività e la correttezza dei lavori. provvedimento incentiverà sicuramente il sistema bancario a tornare ad acquistare crediti, ma possiamo e dobbiamo fare di più. Infatti, il Governo sta studiando una piattaforma che aiuterà le banche a smaltire i crediti acquisiti. Sarà sufficiente? Me lo auguro, ma siamo pronti a sostenere il Governo su altri interventi, purché il problema dei crediti incagliati venga definitivamente risolto.

la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di utilizzare detti crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro; la proroga al 30 settembre del termine per avvalersi della detrazione del 110 per gli interventi realizzati sulle unifamiliari; la remissione *in bonis* destinata ai contribuenti che non rispettano Per le spese sostenute nel 2022 vi è inoltre la possibilità per il contribuente di ripartire la detrazione in dieci quote annuali:

Al fine di salvaguardare i conti pubblici, il decreto blocca il mercato delle cessioni degli sconti in fattura, preservando i lavori in corso. Sono esclusi dal blocco delle cessioni gli interventi per i quali siano stati presentati la Cilas o il titolo abilitativo, gli interventi per i quali non è prevista la presentazione del titolo abilitativo, purché siano iniziati i lavori. Le modifiche alla Camera anche in questo caso hanno escluso dal blocco tutta una serie di interventi di valenza valenza sociale, quali per esempio quelli degli IACP, delle cooperative edilizie, delle ONLUS, nonché gli interventi relativi al superamento delle barriere architettoniche o quelli realizzati nei territori colpiti da eventi sismici o da eventi meteorologici.

ma è stato un *bonus* anomalo, con cui lo Stato non solo ti rimborsa il costo dei lavori, ma ti dà un 10 per cento in più e ti permette di non sborsare in anticipo neanche un euro perché puoi cedere il credito. Non poteva essere sostenuto a lungo. Se aggiungiamo l'alto impatto delle truffe, la lievitazione dei prezzi, le decine di modifiche in corso d'opera che hanno creato confusione e sfiducia, diventa evidente la necessità di intervenire per salvaguardare i conti pubblici tornando alle regole che hanno sostenuto l'economia del settore e aiutato i proprietari di casa per tanti anni. Ricordo che il sistema di pagare gli interventi in anticipo e detrarli in dieci anni ha funzionato splendidamente fin dal 1998 con l'istituzione della e continuerà a funzionare d'ora in avanti, perché vi ricordo che abbiamo fermato la cessione dei crediti, non i *bonus* edilizi. Con i passi avanti fatti nella risoluzione dei problemi legati allo smaltimento dei crediti incagliati e alla messa in sicurezza dei conti pubblici tramite il blocco della cessione si può pensare al futuro. Per espandere la platea di chi accede agli incentivi, per dare stabilità alle imprese è necessario stabilizzare i *bonus* rendendoli pluriennali. Solo così aziende e condomini potranno programmare gli interventi negli anni, dando sicurezza lavorativa al settore dell'edilizia ed evitando quello che io chiamo la rincorsa al ponteggio, che porta al caro materiali e alla conseguente bolla dei prezzi. La stabilità dei *bonus* e la programmazione sono la via per efficientare gli edifici senza correre e senza imporre tempi ai cittadini. È per questo che il Governo e la maggioranza parlamentare non devono abbassare la guardia. Sullo sfondo rimane il grande problema delle case *green* di ispirazione europea: la classe E entro il 2030, la classe D entro dieci anni. Sono obiettivi giusti, ma impossibili da raggiungere nel nostro Paese in tempi così brevi. Siamo un Paese di centri storici impossibili da adeguare; siamo un Paese con tanti condomini in cui non tutti possono affrontare le spese richieste: famiglie che verrebbero costrette dalla maggioranza assembleare ad affrontare spese senza avere disponibilità economica, correndo il rischio di perdere il proprio alloggio. Nomisma ieri alla Camera ha stimato in 350 miliardi il costo per adeguare quasi due milioni di edifici. Quando il Governo Berlusconi abrogò l'IMU

Non lo può fare lo Stato e sicuramente non possono gravare sulle tasche degli italiani. Occorre ribadire all'Europa in maniera ferma che in Italia la casa è sacra, che non vogliamo creare case di serie A e di serie B facendo perdere valore agli immobili delle famiglie meno abbienti che non possono permettersi i lavori di adeguamento. Come ci ha insegnato il presidente Berlusconi - e colgo l'occasione per fargli i miei migliori auguri di pronta guarigione - la casa rappresenta non solo il risparmio degli italiani ottenuto con il sudore di una vita di sacrifici, ma anche le radici di ogni famiglia, l'eredità economica e culturale che ogni padre e madre vuole lasciare ai propri figli. È per questa ragione che annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, perché le disposizioni del decreto-legge in esame percorrono la strada auspicata da Forza Italia e perché siamo orgogliosi di sostenere un Governo che sa risolvere i problemi, anche quando ci sono scelte importanti e difficili da compiere, e sa fare con fermezza gli interessi dei cittadini italiani.

L'economia italiana era totalmente svanita, le imprese erano chiuse, la gente non lavorava; ci siamo trovati a governare forse la fase più difficile dal Dopoguerra in poi. È stato un periodo in cui molti italiani sono stati colpiti sul piano economico, ma anche e soprattutto sul piano umano e sociale. certe parole che dimenticano da cosa è nato il superbonus fa male. C'è molta falsità in quello che ho sentito. Il superbonus è stata una misura geniale, rivoluzionaria e straordinaria, di cui andiamo fieri. Possiamo dire che grazie a questa misura l'Italia è ancora viva. Il superbonus ha consentito in due anni all'Italia, storicamente fanalino di coda dell'Europa, con il PIL più basso per decenni e un'edilizia morta,

per il numero di cittadini. È un calcolo così banale e così falso che veramente porta qualunque forza politica a chiedersi se sia possibile che Giorgetti sia un ministro della Repubblica italiana.

delle ricadute economiche in un periodo difficilissimo e che ha generato quasi un milione di nuovi posti di lavoro. Non bisogna banalizzare una misura che ha avuto degli utili. Perché Giorgetti non ci dice quanta NADEF, quanta cassa integrazione ha evitato il superbonus? Perché non ci dice quanti Comuni hanno incassato dalle sanatorie e quanto incasseranno con la nuova tassa dei rifiuti *(Applausi)*, che aumenta la dimensione delle case e crea una rendita comune grazie alla sanatoria sul superbonus? Allora perché non ci dite non ci dite quante tasse sono entrate in più grazie al superbonus di IVA, Ires, Irap e contributi previdenziali dei 900.000 occupati, che poi hanno fatto probabilmente un mutuo e comprato le case che restauravano? Non si può semplificare una misura economica senza parlare delle interconnessioni economiche che ci sono. I superbonus non sono stati solo costi. Dobbiamo dire ad alta voce che i superbonus sono stati utili. È stata una misura che andava fatta così, in quel periodo storico, perché il Paese era a terra. Il problema è nato quando è finita la pandemia; allora, sì, quella misura andava attualizzata, creandone una di medio e lungo periodo che magari smobilitasse anche dei capitali privati. Ricordiamoci che nel nostro Paese ci sono 1.200 miliardi sui conti correnti. Era giusto quindi poi attualizzare e non correggere quella misura, collega, perché le misure seguono l'andamento della vita e non potevamo prevedere in quel momento quanto sarebbe durata la pandemia. Quindi finché c'è stata la pandemia quella misura andava bene; finita la pandemia, andava non corretta, ma attualizzata alle nuove condizioni del Paese, prevedendo giustamente un *décalage* magari per i redditi più alti; si poteva togliere, per esempio, la batteria ad alcuni interventi, che magari erano meno significativi, e si poteva creare una misura sostenibile nel medio lungo periodo. Non è stato fatto e ciò ha comportato la caduta del Governo Draghi. Lo abbiamo fatto cadere proprio per il superbonus, perché ha bloccato i crediti creando un clima di sfiducia.

e quindi è stata anche una misura rivoluzionaria. Il MoVimento 5 Stelle ha indovinato il settore su cui intervenire, perché l'edilizia muove 18 indotti. Quando facciamo partire l'edilizia lavorano tutti: il piastrellista, l'intonacatore, l'idraulico, l'elettricista. Quindi, abbiamo creato un effetto leva enorme,

per fare degli interventi di efficientamento energetico potrà non piacervi, ma allora cosa proponete? Qual è la vostra visione per raggiungere la direttiva e gli obiettivi che l'Europa ci pone? Se il superbonus non vi piace, diteci voi qual è la misura che voi proponete in alternativa.

Fanno male tutti questi dati falsi e non veritieri, a cominciare da quelli che hanno diffuso il ministro Franco e il governatore Draghi, come l'affermazione che il superbonus era pieno di truffe, scambiando il superbonus con il *bonus* facciate. È grave.

Oggi dobbiamo parlare di come fare a raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci pone ed è possibile; bastava adeguare il superbonus alle nuove condizioni di mercato, lasciando il 100 per cento magari a tutte le case popolari, all'Istituto

Potevamo lasciare la stessa misura al 100 per cento sui redditi bassi e fare un *décalage* sui redditi medi e sui redditi alti per consentire agli investimenti privati di coprire quell'eccesso, magari pagato dallo Stato, e tutto ciò anche se i conti non li abbiamo perché - come vi ho detto - c'è chi dice anche che il superbonus ha prodotto di più di quello che è costato, e quindi dobbiamo partire dai dati. Sul superbonus servono dati seri e certi per creare una misura analoga che riesca magari a far intervenire anche il capitale privato e ci possa far raggiungere gli obiettivi che l'Unione europea ci chiede. Anche perché la scorsa settimana, o dieci giorni fa, o dieci giorni fa, una madre ha lasciato orfano un bambino proprio per un'esplosione di gas e quindi dobbiamo elettrificare le nostre abitazioni. Dobbiamo ridurre l'inquinamento: ogni anno ci sono 70.000 morti per l'inquinamento nelle città e questo può succedere a tutti noi. Dobbiamo dunque andare in quella direzione e quindi un fisco piatto piatto e insignificante non ha senso. A noi serve un fisico che premi coloro che vogliono fare interventi *green* e a coloro che faranno interventi *green* abbasseremo le tasse. Dove purtroppo non c'è capienza fiscale, dovrà essere lo Stato ad intervenire, in modo da consentire a tutti di poter vivere in un ambiente sicuro e sano. Concludendo: di cantieri ne ho visitati e da ne ho visitati e da quando c'è il superbonus abbiamo avuto più sicurezza nei cantieri e zero sommerso, perché le imprese assumevano a tempo indeterminato.

Allora continuate su questa strada! Vedo che qualcuno annuisce. Ecco perché il nostro voto è fortemente contrario e aspettiamo dal Governo una visione che possa indirizzare il nostro Paese verso l'innovazione, il cambiamento e una modernizzazione che ormai non può più aspettare.

secondo luogo, sentendo qualche intervento di chi mi ha preceduto, in particolare l'ultimo, sembra quasi che questo intervento del Governo sia il problema, quando invece è la soluzione. *(Applausi)*. Cerchiamo di fare ordine: se andava così bene, con queste norme, come mai ci sono stati miliardi di euro Come mai ci sono stati e ci sono ancora quasi 20 miliardi di euro di crediti incagliati, che poi è un brutto termine per dire che ci sono aziende che hanno lavorato e fanno fatica a recuperare i soldi? Se tutto fosse stato così perfetto, stati questi problemi. Evidentemente non era così perfetto ed era necessario intervenire. Il Governo è intervenuto e ringrazio il ministro Giorgetti, il presidente Meloni e tutto il Governo, perché lo ha fatto con buon senso,

parte del caos nasce dalle prime norme, che non prevedevano certificazioni. Non ci fosse stata la stretta fatta a novembre 2021 dal Governo Draghi, sarebbe successo un putiferio. Quindi le norme erano scritte male e hanno consentito errori che adesso dobbiamo risolvere. È compito di tutti, non della maggioranza o dell'opposizione, ma è compito del Parlamento. Noi siamo la fabbrica delle leggi e abbiamo il dovere di risolvere i problemi. Quindi ci si dice che, giustamente, con il 110 per cento, la cessione del credito e lo sconto in fattura l'economia è ripartita. Bella forza! Se si mettono 120 miliardi di euro nell'economia, è ovvio che l'economia riparte. Non ci vuole uno scienziato in economia per capire che, mettendo 120 miliardi di euro, il PIL cresce. Il punto è come, se cresce senza evitare distorsioni, truffe e inflazione. Il nostro dovere infatti è fare le cose bene: non perfette, perché è impossibile, però almeno decentemente bene. Dunque cerchiamo di capire

Certo, per anni la Guardia di finanza girerà col trapano per vedere se c'è il cappotto o no quanto è profondo, se corrisponde a quanto dichiarato o no. Quindi per anni la Guardia di finanza andrà a riprendere le teste di legno che hanno dichiarato il falso. Ahimè, sarà difficile recuperare quello che è stato monetizzato, quello che è volato all'estero in paradisi fiscali. Quindi il tema chiaro è che va bene la buona fede, però le norme erano fatte male.

ma la vecchietta che deve rifare il bagno e non accede al superbonus, la caldaia la paga il doppio, le piastrelle le paga il doppio. Paga tutto il doppio. una norma fatta in buona fede, ma male, ha creato una distorsione del mercato e inflazione che pagano - guarda caso - le persone con meno risorse. Andiamo poi a vedere il carattere regressivo del per cento. Capisco benissimo, infatti, e poi lo dirò in conclusione, che è giusto che il Governo prosegua nell'aiutare le fasce deboli, gli IACP e le case popolari, ci mancherebbe altro, però il problema è che, per come è nato, ha favorito soprattutto i ricchi. Le seconde case non le hanno i poveretti. Aveva senso farlo per le seconde case? Questa cosa, onestamente, non l'abbiamo mai capita,

regalato la ristrutturazione a persone abbienti. Non è il massimo dell'efficienza. Ma veniamo alla fine: ci si dice, giustamente, una serie di misure fatte in un momento di difficoltà, il che è verissimo, che hanno fatto ripartire l'economia, ed è vero, lo abbiamo detto prima che se investi 120 miliardi l'economia riparte. Banca d'Italia, però, ha smontato il mito del moltiplicatore al mille per mille: è meno dell'uno. Quindi è un moltiplicatore inferiore a uno. Stanziati 120 miliardi, va bene se ne tornano 100. Questa è la prima parte del problema. La seconda parte del problema è Eurostat che

io sarò all'antica, ma come funziona il bilancio dello Stato? Cerchiamo di farlo capire anche a chi non se ne occupa. Il bilancio dello Stato è facilissimo: ci sono entrate e uscite. Se le entrate sono inferiori alle uscite, stai spendendo di più di quello che entra. E secondo voi, come si paga la differenza? Con il

Dunque, ha fatto benissimo il Governo a imporre una stretta immediata, perché altrimenti quest'anno avremmo avuto un'esplosione di *deficit*, non coperta e che avremmo dovuto coprire con tasse. conclusione, perché quello che c'era da dire lo abbiamo detto, il Governo ha preso una ottima iniziativa, di buon senso, con una uscita *soft*, non da misure sbagliate in quanto tali, ma da misure scritte male.

il Gruppo del Partito Democratico voterà contro la questione di fiducia posta a nome del Governo dal ministro Ciriani. Per noi ci sono ragioni di metodo e ragioni di merito, il collega Fina ha ben argomentato nel suo intervento. Io voglio partire dal metodo. Noi ormai riteniamo insostenibile proseguire senza aprire in Parlamento il cantiere delle riforme, con un monocameralismo improvvisato, che in una democrazia parlamentare sottrae ad un ramo del Parlamento la possibilità di esprimersi e di raccogliere le istanze dei cittadini e delle imprese. Il problema, lo sappiamo, non nasce in questa legislatura. Tuttavia, l'Italia è fuori dall'emergenza pandemica. Con le elezioni politiche si è insediata una maggioranza. La stessa si definisce legittimata dal voto dei cittadini. È certamente legittimata nell'importante esercizio di governo, ma non è legittimata ad accompagnare su un piano inclinato le nostre istituzioni democratiche, violando l'impianto costituzionale. Signor Presidente, dobbiamo ridefinire metodi e tempi con i quali il Governo definisce e approva i decreti-legge. Serve una nuova programmazione, perché questi decreti troppo spesso restano alcuni mesi in un ramo del Parlamento, per poi divenire veicoli *omnibus* su temi e materie in molti casi lontani dalle prerogative della decretazione. Sul merito, il senatore Garavaglia cerca di rappresentare il decreto-legge come la soluzione alla questione della cessione dei crediti. in punta di piedi e con grande equilibrio, vorrei ricordare al senatore Garavaglia che se fosse così, se il Governo avesse risolto la questione della cessione dei crediti, non ci sarebbero decine di migliaia di imprese centinaia di milioni di lavoratori che in questo momento stanno protestando, perché a rischio ci sono i cantieri, il lavoro e la tenuta di decine di migliaia di imprese nel nostro Paese. Peraltro, le numerose modifiche introdotte alla Camera dei deputati evidenziano le grandi lacune con le quali è stato approvato dal Consiglio dei ministri questo decreto. Un decreto in molti casi confuso, senza una chiara prospettiva, soprattutto carente di un impianto che, a mio avviso, dovrebbe tener conto della importante missione che gli interventi, pubblici e privati, hanno nella definizione della crescita del nostro Paese. Abbiamo ridotto il danno anche grazie a tante nostre proposte: la reintroduzione della cessione del credito per le case popolari e per il terzo settore; le agevolazioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche; gli interventi correttivi introdotti a tempo scaduto sulle aree terremotate e alluvionate. Non tenerne conto in un decreto d'urgenza con il quale il Governo interviene, mostra un problema strutturale: manca in questo decreto una visione, un progetto, una prospettiva. Lo abbiamo più volte ricordato: qui ci sono 19 miliardi già maturati che mettono a rischio 115.000 cantieri, 32.000 imprese, 170.000 lavoratori. Voglio domandare al Governo, attraverso la Presidente: come intendete salvaguardare il lavoro e l'impresa? Continuo a pensare che su questa domanda così importante ci siano confusioni, soluzioni inappropriate e inadeguate, sottovalutazioni di questioni fondamentali. Un grande Paese manifatturiero, la seconda manifattura (perché questo rappresenta il nostro Paese), non può permettersi un Governo che si limita ad un'opposizione al passato, anziché guardare al presente e al futuro dell'economia e della società italiana. Abbiamo un bisogno urgente, ad esempio sugli investimenti pubblici e privati, di abbracciare il futuro. La transizione in chiave ecologica della nostra economia, sia essa energetica, digitale o sociale, richiede un progetto, un testo unico. Lo diciamo al Governo: aprire il cantiere della definizione di un testo unico per sostenere gli investimenti pubblici e privati richiede sull'efficientamento energetico una progettualità, non l'individuazione di un colpevole in una direttiva europea, che peraltro segna un passo in avanti, non un passo indietro. Per quale ragione non avete accompagnato a questo decreto-legge una proposta, un testo unico di riorganizzazione dei *bonus* in edilizia? L'esigenza di efficientare ambientalmente i nostri fabbricati e di consolidare la tenuta statica degli stessi è tuttora una priorità, per non dire un'emergenza, in un Paese che ha un patrimonio edilizio peraltro in molti casi datato e incompatibile con l'esigenza che abbiamo di ridurre le emissioni, di non consumare materie prime, che peraltro in molti casi sono limitate. Senza un progetto, senza una visione, senza una nuova progettualità, non basta l'individuazione dei costi. 110 era una misura nata durante una pandemia, utile a rimettere in cammino il Paese; sapevamo che era costosa e che non poteva divenire strutturale; ma sapevamo altresì con grande chiarezza che da un Governo e da una maggioranza politica legittimata dal voto ci si attende una proposta, non un'accusa al passato. Mi chiedo e lo hanno ricordato molti colleghi: come si pensa di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza se si lasciano le imprese delle costruzioni nelle procedure fallimentari? Guardate che quando chiude un'impresa o quando un'impresa entra in procedure fallimentari non riesce più a partecipare ai bandi di gara. Le stazioni appaltanti vanno deserte negli appalti fondamentali per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qui ci si gioca l'Alta velocità, non un contributo - tanto per essere chiari - dato ad un privato, senza una visione economica su come mettere in sicurezza un comparto delle costruzioni che peraltro negli ultimi anni ha anche fatto numerosi investimenti. Quali sono le politiche economiche che avete in testa per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, se si lasciano 30.000 imprese dentro possibili procedure fallimentari? Ma come faremo mai ad accompagnare un progetto di crescita, di innovazione, di prospettiva nel nostro Paese? Questa è la questione politica che noi poniamo. Ecco perché diciamo che in gioco c'è il destino di un pezzo dell'economia italiana. Non ho bisogno qui di ricordare cosa rappresenta il comparto delle costruzioni, in un'alleanza tra lo Stato e il mercato per creare un processo di crescita socialmente sostenibile Il Governo non sta facendo i conti per verificare quanto costerebbe, in termini di ammortizzatori sociali, lasciare nelle procedure fallimentari migliaia di imprese in questo Paese, alla vigilia di un Piano nazionale di ripresa e resilienza tuttora confuso,

le funzioni fondamentali. È l'asse fondamentale della crescita e dello sviluppo economico che questa maggioranza ancora non è in grado di rappresentare in quest'Aula. Ecco perché riteniamo, collega Garavaglia, - lo dico con grande rispetto - che non si possa definire questo decreto-legge risolutivo dei problemi della cessione del credito, perché questo decreto-legge manca di quella prospettiva fondamentale che ho richiamato poco fa, quella di un'idea dello sviluppo economico e sociale di questo Paese. Io penso che sui bonus edilizi serva un testo unico, perché vorrei raggiungere obiettivi più sfidanti in termini di riduzione delle emissioni e in termini di consolidamento. Quanto ci costa, ad esempio, rincorrere sempre in emergenza il dissesto idrogeologico? Quanto spendiamo per finanziare commissari ed emergenze che segnano l'assenza di una procedura di manutenzione e di sostegno che il pubblico deve avere nei confronti del nostro Paese? Queste sono le ragioni di metodo e di merito che richiedono l'apertura di un cantiere nuovo da parte di questa maggioranza. Venite via dall'idea che sia sufficiente governare un grande Paese facendo opposizione al passato. Entrate nell'ottica che su di voi c'è una responsabilità di Governo, c'è la responsabilità di indirizzare nel futuro questo Paese. Lo dico perché produrre occupazione di qualità, produrre sviluppo economico e produrre crescita non è un esercizio che che può limitarsi a un'accusa al passato, ma è un faticoso esercizio che richiede un'idea dello sviluppo economico. Lo dobbiamo prima di tutto alle giovani generazioni.

nulla di scritto, perché in questi mesi abbiamo lavorato in Commissione su una serie di problemi. Tutti i Governi ereditano problemi e tutti i Governi si candidano. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un Governo politico, con una propria *Weltanschaung* Penso che sia giusto ricordare a voi, cari colleghi della minoranza e dell'opposizione, che ci sono alcune cose che in questi anni dovremo fare insieme. C'è uno Stato, al di là della pandemia e al di là di una guerra che nessuno poteva immaginare, figuratevi noi che per la prima volta, dopo una traversata nel deserto, ci troviamo con la responsabilità di governare questo Paese e questa Nazione. C'è un'idea complessiva, che penso debba appartenerci: l'idea che questo Stato organizzato a livello orizzontale e verticale non funziona, l'idea che, rispetto a questo Stato, sia necessario dare una

con circa di 41 soggetti che a vario titolo si sono occupati dei diversi crediti di imposta e delle cosiddette spese fiscali di questo Paese che vanno riformate. Questo tema si inserisce in una visione complessiva

Non lo ha scritto Conte, non lo avete scritto voi perché gli altri provvedimenti avevano tutti una grande fantasia: desidero ricordare i banchi a rotelle, insomma tante altre cose fantasiose. Abbiamo visto la fantasia al potere, quindi mi rivolgo soprattutto ai colleghi del PD, a chi deve dare a questo Paese due diverse visioni del mondo, quella conservatrice e quella progressista o come le volete definire, una stabilità di confronto. Sappiamo che la vostra visione del mondo è stata per tanti anni minoritaria in questo Paese, tanto che

significa avere al Governo, per la prima volta nella storia di questo Paese, chi guarda l'Italia con unitarietà e sceglie anche di accettare la sfida di un regionalismo differenziato, perché francamente per cinquant'anni, per me che vengo dalla Calabria, non abbiamo trovato tutte queste soluzioni. Si abbia il coraggio di dire insieme

Questo non è un provvedimento rivoluzionario, è ben altra la rivoluzione che noi immaginiamo. Questo è un provvedimento che, speriamo insieme, coglie i limiti

rispetto a chi non comprende il valore della storia, posso dire che sono nato nel 1971; mio nonno faceva l'elettricista e sono davvero nauseato da questo racconto di chi, è portatore di una sensibilità politica minoritaria nel Paese, ogni volta deve aggredire e pensare noi siamo nostalgici non so di quale storia. Io so che noi siamo nostalgici magari, che so, di Leon Battista Alberti; in alcuni tempi finanche gli statunitensi venivano a studiare quella visione a quella architettura che ci ha consegnato piazze e paesi *(Applausi)*. Altri invece che hanno governato ci hanno consegnato con il consenso del Parlamento e

noi abbiamo nostalgia di chi si occupa di questo Paese con grande orgoglio, con chi pensa al merito. In tutti questi provvedimenti, anche in quello che stiamo discutendo, che va a risolvere i problemi

ai colleghi del PD e di Azione, alla collega Paita. Condivido l'idea che una visione strutturale, come stiamo facendo in Commissione, una tassazione che stava lì dal 1973, possa restituire una nuova visione economica dell'Italia, possa restituire investimenti con blocchi, come sempre è stato.

a parlare lo smacchiatore di giaguari, che addirittura ci dice che siamo fuori dall'arco costituzionale. Non so, e addirittura ci dice che Berlusconi e l'UDC hanno palleggiato, fosse quasi una minaccia. Penso che a lui, a questo Parlamento, ai nostri figli che stanno a casa, noi nel tenere unito questo Paese, che vive dei principi costituzionali, non dobbiamo dimostrare - ripeto né a smacchiatori di giaguari né a qualcun altro - di essere aderenti alla Costituzione. Magari qualcuno vorrebbe che cantassimo «Bella ciao». Continueremo invece a servire le istituzioni e i momenti istituzionali. Sarà così anche per il 25 aprile, annunciato dal presidente Meloni e dal presidente La Russa. Perdonateci rispetto a una canzone che ha poco *groove*, continueremo con il sorriso, magari continuando a cantare Battisti, mentre anche oggi in Parlamento esprimiamo un voto favorevole su un provvedimento importante del Governo che risolve un problema.

con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.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 luogo mediante votazione nominale con appello. Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no;

Malan

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,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

Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche giorno fa poteva essere mio figlio a trovarsi presso una pompa di benzina a San Giovanni a Teduccio e non quell'ingegnere raggiunto da due colpi di pistola per essersi opposto ai rapinatori che volevano rubargli lo *scooter;* magari poteva essere mia figlia a trovarsi lungo la traiettoria di un colpo partito dalla pistola di un diciannovenne nell'affollatissima zona di Mergellina, com'è accaduto a Francesco Pio, quando un suo coetaneo, che aveva subito il disonore di un pestaggio di scarpe, con metodo mafioso ha estratto la pistola, sparando per intimidire ad altezza uomo, ferendo a morte un diciottenne. Chiediamoci perché un giovane debba uscire con una pistola in tasca in piena *movida.* Onorevoli colleghi, i miei figli, per diversi motivi che solo il fato serba in grembo, potevano trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma chi si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, quando i colpi di pistola trafiggono vittime innocenti? Cosa c'è di sbagliato nel camminare lungo la strada col proprio figlio, come faceva Silvia Ruotolo, quando fu freddata dalla camorra per sbaglio? Cosa c'è di sbagliato nel camminare per strada, come stava facendo la piccola Annalisa Durante, che si trovò lungo la traiettoria di una sparatoria? Cosa c'è di sbagliato nello stare seduto su una panchina, come Genny Cesarano, ucciso per errore durante una stesa? Sempre e solo i criminali si troveranno dalla parte sbagliata della storia, ma a che serve condannare, se dalle parole non si passa ai fatti? confermano che ancora oggi la città di Napoli è preda della criminalità e di un forte disagio sociale che verrà alimentato ancor di più da provvedimenti che porteranno a delinquere chi non riesce nemmeno a mettere il piatto a tavola, come l'abolizione del reddito di cittadinanza. Onorevoli colleghi, magari domani possiamo riflettere sulle misure da mettere in campo per staccare la spina alla piaga della criminalità, per colmare il vuoto educativo e culturale, per creare occupazione e soprattutto per sostenere e rafforzare la scuola di ogni ordine e grado, che sia gratuita, a tempo pieno e aperta al territorio. Oggi però la gente muore. Oggi questo Governo deve dare risposte rapide e concrete alla mia terra, dispiegando uomini, fondi e mezzi e ascoltando il grido di dolore che si leva dalle nostre Forze dell'ordine, in perenne sottorganico e senza nemmeno le risorse per la benzina. Onorevoli colleghi, per rinnovare il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, il mio popolo non chiede privilegi, ma solamente il rispetto di quegli stessi diritti garantiti in altre parti del Paese. Spero di non parlare a vuoto, considerando che l'autonomia differenziata non potrà che acutizzare la sperequazione dei diritti a danno dei territori più fragili.

la notte tra il 5 e il 6 aprile volarono in cielo 309 vittime *(Applausi)*, amici, parenti, compaesani e concittadini che non ci sono più; non sono più con noi, ma vivono nel ricordo che quotidianamente noi, che abbiamo vissuto da vicino la tragedia, ma anche tutti gli italiani, e non solo,

nel 2009 ha purtroppo manifestato tutta la sua forza distruttiva. Dal terremoto del 1700 i colori della città de L'Aquila, che erano il bianco e il rosso, sono diventati il nero e il verde, gloriosi colori oggi,

di *mea culpa* per gli errori che abbiamo commesso in passato, dai quali stiamo imparando nel tempo per quanto riguarda la ricostruzione, per mettere a posto il nostro tessuto

in difficoltà e stavamo riflettendo su cosa dovessimo fare, se votare qui la fiducia o andare all'Aquila, dove in questo momento è in corso una cerimonia religiosa in ricordo delle 309 vittime del terremoto. Il Presidente del Consiglio e metà Governo

Abbiamo però deciso di essere qui perché questo è quello che i nostri concittadini ci hanno chiesto: i nostri concittadini hanno voluto che votassimo votassimo provvedimenti come quello relativo al *bonus* e, in particolar modo, nell'ambito di questo decreto, al sismabonus, che sarà importantissimo per portare avanti la ricostruzione di quello che ancora non è stato ricostruito. Sarà importante spostare tutto quello che di buono abbiamo partorito nel 2009 in termini di ricostruzione anche sui crateri successivi, come quello, in particolar modo, del Centro Italia.

sceglie per immedesimarsi in tutto quello che abbiamo passato in quei momenti. Non lo auguriamo a nessuno, ma oggi è anche un momento, per quanto mi riguarda, per guardare lontano e con positività ai prossimi anni e alla possibilità

fornirono alla città dell'Aquila - che giunse anche da questi banchi, tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza, perché i Governi che si sono succeduti hanno dato tutti testimonianza di forte attaccamento alla tematica - è il vero segno di quanto questa Nazione sia la migliore del mondo. Grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che faremo tutti quanti insieme.